Onorevoli senatori, l'età avanzata, sotto altri aspetti aggravante, mi conferisce oggi l'incarico di presiedere l'inizio della XVI legislatura del Senato della Repubblica, nel quale, sessant'anni or sono, ebbi il privilegio di assistere come Sottosegretario alla prima seduta. Doveroso e sentito è l'omaggio al Capo dello Stato

insieme al saluto augurale ai nuovi appartenenti a questo ramo del Parlamento e a quanti hanno già avuto, qui o alla Camera, lo stesso altissimo mandato. Usa sempre dirsi che si passano momenti difficili, ed è appropriato, ma tutte le difficoltà sono adeguatamente affrontabili e superabili se i rappresentanti del popolo sanno interpretare puntualmente aspirazioni ed esigenze, trovando possibili rimedi. Aggiungo soltanto una parola,

che presiedette splendidamente il Senato, interpretandone doveri e diritti.

BONINO. Chiedo la parola per un richiamo al Regolamento, a norma dell'articolo 4 del Regolamento del Senato, e per porre conseguentemente la mia candidatura alla Presidenza del Senato. Da trent'anni noi riteniamo che queste candidature vadano parlamentarizzate: non si sentono dall'ANSA o dai giornali, non si discutono nei caminetti. Per questo motivo - signor Presidente, la ringrazio pongo la mia candidatura alla Presidenza del Senato. secondo la quale la nostra Assemblea opera in questa fase esclusivamente come seggio elettorale. Essa non può Essa non può adempiere ad incombenze diverse da quelle tassativamente elencate dal suddetto articolo. Per questi motivi, anche in conformità ad una prassi consolidata, non sono ammessi interventi per la presentazione di candidature o discussioni delle stesse, come non sono ammesse dichiarazioni di voto. Le richieste avanzate in tal senso non possono quindi essere accolte. L'elenco dei senatori in congedo sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta Comunico che, in data 24 aprile 2008, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo»

L'ordine del giorno reca: «Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio». A norma dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, invito i senatori Massimo Garavaglia, Anna Rita Fioroni, Donatella Poretti, Enrico Montani, Marco Perduca e Simona Vicari, che risultano essere i più giovani senatori presenti in Aula, a prendere posto al banco della Presidenza per esercitare le funzioni di Segretari provvisori. Comunico che i senatori Astore, Belisario, Calderoli, Castelli, Finocchiaro, Mariapia Garavaglia, Latorre e Marini, proclamati eletti per il Senato in più Regioni, hanno indicato le loro rispettive opzioni: il senatore Giuseppe Astore, eletto per la lista «Italia dei valori-Lista Di Pietro» nelle Regioni Lombardia e Molise, ha dichiarato di optare per la Regione Molise; il senatore Felice Belisario, eletto per la lista «Italia dei valori-Lista Di Pietro» nelle Regioni Puglia e Basilicata, ha dichiarato di optare per la Regione Basilicata; il senatore Roberto Roberto Calderoli, eletto per la lista «Lega Nord» nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Friuli-Venzia Giulia, ha dichiarato di optare per la Regione Lombardia; il senatore Roberto Castelli, eletto per la lista «Lega Nord» nelle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, ha dichiarato di optare per la Regione Liguria; la senatrice Anna Finocchiaro, eletta per la lista «Partito Democratico» nelle Regioni Emilia-Romagna e Lazio, ha dichiarato di optare per la Regione Emilia-Romagna; la senatrice Mariapia Garavaglia, eletta per la lista «Partito Democratico» nelle Regioni Veneto e Lazio, ha dichiarato di optare per la Regione Veneto; il senatore Nicola Latorre, eletto per la lista "Partito Democratico" nelle Regioni Puglia e Basilicata, ha dichiarato di optare per la Regione Puglia; senatore Franco Marini, eletto per la lista "Partito Democratico" nelle Regioni Lazio e Abruzzo, ha dichiarato di optare per la Regione Abruzzo. Comunico che, in data 28 aprile 2008, è pervenuta al Presidente una lettera con la quale il senatore Galan Galan dichiara di dimettersi dalla carica di senatore, al fine di proseguire il proprio mandato di Presidente della Regione Veneto. Trattandosi di dimissioni motivate da incompatibilità, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, l'Assemblea non può che prenderne atto. finestra"). L'ordine del giorno reca: «Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti». La Giunta ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati che subentrano agli optanti per altre circoscrizioni e al senatore dimissionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento, la Giunta provvisoria è costituita dai senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica della precedente legislatura che sono presenti nella seduta, in numero non inferiore a sette. Invito, pertanto, i senatori Alberti Casellati, Augello, Berselli, Carloni, Carrara, Casson, Giuliano, Legnini, Lusi, Malan, Nania, Negri e Pastore a riunirsi immediatamente nell'adiacente sala Pannini per procedere a tali accertamenti. Per consentire alla Giunta provvisoria di adempiere ai propri compiti, sospendo la seduta, che riprenderà non appena tali lavori saranno conclusi. *(La seduta, sospesa

alle ore 10,56).* Comunico che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri ha concluso i propri lavori. Invito pertanto il senatore Segretario provvisorio a dare lettura della proclamazione dei candidati che risultano primi dei non eletti nei seggi resisi vacanti. Informo che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri ha comunicato di aver preso atto delle dichiarazioni di opzione pervenute e, per le sostituzioni cui occorre provvedere nei seggi resisi in conseguenza vacanti, ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale per il Senato, ha riscontrato che nelle sottoindicate Regioni risultano primi dei non eletti i seguenti candidati: nella Regione Piemonte, per la lista "Lega Nord", Rossana Lidia Boldi, in sostituzione del senatore Roberto Calderoli; nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per la lista "Lega Nord", Mario Pittoni, in sostituzione del senatore Roberto Calderoli; nella Regione Lombardia, per la lista "Di Pietro-Italia dei valori", Gianpiero De Toni, in sostituzione del senatore Giuseppe Astore e, per la lista "Lega Nord", Irene Aderenti in sostituzione del senatore Roberto Castelli; nella Regione Basilicata, per la lista "Partito Democratico", Maria Antezza Papapietro, in sostituzione del senatore Nicola Latorre; nella Regione Lazio, per la lista "Partito Democratico", Vincenzo Maria Vita in sostituzione del senatore Franco Marini, Maria Francesca Marinaro in sostituzione della senatrice Anna Maria Paola Luigia Finocchiaro, Roberto Di Giovan Paolo in sostituzione della senatrice Mariapia Garavaglia; nella Regione Emilia-Romagna, per la lista "Lega Nord", Angela Maraventano, in sostituzione del senatore Roberto Castelli; nella Regione Puglia, per la lista "Di Pietro-Italia dei valori", Giuseppe Caforio, in sostituzione del senatore Felice Belisario. Do atto alla Giunta di queste sue comunicazioni e proclamo quindi senatori i candidati Rossana Lidia Boldi, nella Regione Piemonte, Mario Pittoni, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, Gianpiero De Toni e Irene Aderenti nella Regione Lombardia, Maria Antezza, nella Regione Basilicata, Vincenzo Maria Vita, Maria Francesca Marinaro, Roberto Di Giovan Paolo, nella Regione Lazio,

altresì che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto, a seguito delle dimissioni del senatore Giancarlo Galan, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Piero Longo. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Piero Longo. Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ricordo che in questo scrutinio per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, e cioè 162 voti. Per garantire un ordinato svolgimento delle operazioni di voto, come è avvenuto per l'elezione del Presidente nella passata legislatura, davanti al banco della Presidenza è stata approntata una cabina. I colleghi senatori, prima di entrarvi, riceveranno dagli assistenti parlamentari una scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa. I senatori a vita saranno chiamati per primi ad esprimere il proprio voto. La chiama proseguirà con gli altri senatori in ordine alfabetico.

Di Giovan Paolo,

Onorevoli senatrici, onorevoli senatori, l'alta responsabilità che avete voluto affidarmi mi onora e mi emoziona profondamente. Voglio per questo porgere un sentito ringraziamento a tutti voi. Desidero in primo luogo rivolgere, a nome dell'Assemblea dei senatori e mio personale, un saluto deferente al Capo dello Stato, presidente Giorgio Napolitano supremo garante della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. Le sue doti di saggezza e la sua ferma cultura istituzionale sapranno essere, come lo sono state, una guida ed un valore. Un saluto particolare rivolgo ai Presidenti emeriti della Repubblica ed ai senatori a vita. Permettetemi altresì di esprimere anche il mio ringraziamento al presidente Marini. *(Vivi, In questi anni ho potuto apprezzarne le doti di equilibrio e la capacità di includere in un comune percorso tutte le componenti parlamentari, nella consapevolezza che di questa condivisa partecipazione e non già dell'opposizione sterile e preconcetta la democrazia si nutre. Questo riconoscimento è frutto della mia esperienza di Presidente di un Gruppo di opposizione nella precedente legislatura, durante la quale ne ho più volte dato atto. Così come non posso dimenticare la correttezza e la compostezza del mio confronto con il Capogruppo di maggioranza, senatrice Anna Finocchiaro *(Generali applausi)*, con la quale ho avuto sempre un confronto corretto. Mi preme sottolineare quanto senta alta la responsabilità del ruolo che da questo momento assumo e gli anni trascorsi in quest'Aula mi hanno insegnato quanta sensibilità occorra per guidare i lavori del Senato della Repubblica. Si avvia una gestione che nelle aspettative appare densa di obiettivi da raggiungere, aspettative sulle quali il Senato dovrà impegnarsi perché i risultati corrispondano alle esigenze del Paese. Quanto al mio compito, io mi impegno ad adempierlo con il massimo scrupolo di garante delle regole, dei diritti dell'opposizione, della maggioranza e delle esigenze del Governo. Essere il garante sarà la missione principale da me più volte sentita in questa funzione. So che dovrò assumere le ragioni di tutti e prima ancora il bene supremo dell'Assise che sono chiamato a presiedere, nella piena consapevolezza che dal concorso di tutti e nella salvaguardia di ruoli e posizioni politiche, etiche ed ideologiche dovrà avere luogo anche la necessaria riscrittura delle regole. Questo sarà uno degli elementi fondanti di questa legislatura che si apre, durante la quale è indispensabile che si sappia conservare e preservare il valore della reciproca legittimazione delle parti emerso sul finire della scorsa legislatura in occasione dell'apertura del dialogo sulla legge elettorale. Questa reciproca legittimazione rafforza il Parlamento, consente a maggioranza e opposizione di operare per l'ottenimento del bene più importante, cioè la crescita del nostro Paese e l'affermazione dei valori della Costituzione repubblicana di cui quest'anno abbiamo celebrato il sessantesimo anniversario della sua entrata in vigore. In quella Carta c'è la nostra storia, il nostro passato, le nostre speranze, il nostro futuro. C'è il dolore di una guerra atroce e c'è la rinascita dalle macerie che ha spinto le generazioni che ci hanno preceduto a ricostruire mattone per mattone, pezzo per pezzo, il nostro Paese. E c'è anche la tensione costante da tenere verso il nostro valore più alto e più sacro: la libertà. È questo che ci rende uguali alle grandi democrazie, dove la contrapposizione fra differenti aree politiche, avversarie ma non nemiche, consente ai cittadini di credere che nelle scelte riformiste, di cui anche nel nostro Paese si avverte oggi la necessità, la politica sappia ritrovare la necessaria maturità. L'avvenuta semplificazione del quadro politico potrà aiutare la stabilità e potrà aprire, in tempi brevi, una feconda stagione di riforme condivise. La riduzione dei Gruppi parlamentari potrà rappresentare una significativa facilitazione dei lavori di quest'Aula e delle Commissioni. Quella maturità dovrà essere la fonte primaria per alimentare la capacità di ascolto che le forze politiche oggi rappresentate in Parlamento dovranno esercitare per farsi interpreti di tutte le esigenze del Paese, comprese quelle delle minoranze oggi non più presenti. Questo per la politica è un valore ed è uno degli elementi idonei a ricollocarla al suo posto ambito: non a destra al centro o a sinistra, ma in alto, dove al di là delle democratiche competizioni elettorali e dei suoi esiti è possibile confrontarsi, ciascuno con la propria sensibilità, per il bene comune. Questa semplificazione ne richiama un'altra: quella del linguaggio, della comunicazione politica con la quale il Palazzo non deve più parlare a sé stesso e per sé stesso, ma ai cittadini. Questo attuale tempo della politica ci offre una straordinaria opportunità. Sta a noi coglierla. Quella che ci aspetta sarà la stagione delle riforme, ma anche dell'affermazione della legalità come valore irrinunciabile. Legalità e sicurezza sono le richieste più pressanti che vengono dalla gente, dal Nord al Sud. Insieme infatti all'azione di contrasto a tutte le mafie, occorre intensificare e migliorare le strategie per combattere quella dilagante criminalità che sta rendendo invivibili ampie aree del nostro Paese. Si tratta di un problema che va affrontato con la necessaria attenzione, perché serie e fondate sono le preoccupazioni dei cittadini anche in ordine alla relazione tra una parte significativa dei reati commessi e l'immigrazione clandestina di soggetti con pesanti storie criminali. Abbiamo il dovere, pertanto, di non sottovalutare questi aspetti, agendo con rigore e severità ove occorre, senza dimenticare la grande tradizione di tolleranza e accoglienza che dobbiamo conservare nei confronti di quella immigrazione sana e regolare che ha, invece, bisogno del nostro aiuto. Sono inoltre fermamente convinto che la lotta a tutte le mafie non dovrà avere, ma neanche mostrare, alcuna pausa. Su questo fronte il Parlamento ha legiferato proficuamente, stabilizzando il 41-*bis* (il cosiddetto carcere duro) ed ha sostenuto magistratura e polizia giudiziaria in quella fruttuosa opera che da sette anni ad oggi ha consentito la cattura di pericolosi latitanti ai vertici della criminalità organizzata, recidendo molti rami della mala pianta del *racket* delle estorsioni. Permettetemi di soffermarmi su questo punto. Da siciliano, infatti, sento forte la necessità di un impegno crescente per la sicurezza e per l'affermazione dei valori di legalità perché ho vissuto, insieme a tutti gli altri siciliani, il dolore di vedere la mia terra ferita, vessata, umiliata e, insieme, l'orgoglio di vedere una Sicilia che non s'è mai piegata né mai data per vinta e che è stata capace, invece, di rialzarsi e gridare il suo rifiuto alla violenza, alla prepotenza, all'illegalità. È di grande conforto vedere come nella società emergano e si moltiplichino le scelte virtuose e coraggiose di cittadini e categorie che, a viso aperto, si oppongono alle vessazioni della criminalità organizzata. Ma non è solo sulla necessità di una maggiore sicurezza che Nord e Sud del nostro Paese ci chiedono un forte impegno. L'esistenza di una questione meridionale e di una questione settentrionale appare ormai acclarata, pur nella differenza tra le due aree del Paese, e richiede interventi importanti per superare il divario tra Nord e Sud e per consentire di proseguire un percorso virtuoso di crescita che sia contestuale, se non vogliamo un Paese a due velocità. Il settentrione ha confermato di essere il cuore produttivo del Paese, crescendo nell'efficienza del sistema, integrandosi agli *standard* europei, ma mostrando un crescente bisogno di maggiore efficienza dello Stato e della pubblica amministrazione. Il Mezzogiorno, dal canto suo, ha dimostrato in questi anni di saper trovare la capacità di promuovere uno sviluppo fondato sulle proprie risorse, rifiutando l'assistenzialismo, le prebende e pretendendo invece interventi in favore delle infrastrutture e delle imprese. Soltanto conciliando le esigenze e rispondendo alle istanze delle due aree del nostro Paese, ed impegnandoci con forza e convinzione per tessere quell'indispensabile legame forte tra Nord e Sud, sapremo onorare quell'unità d'Italia così fortemente voluta e di cui, durante questa legislatura che ci si apre, nel 2011 celebreremo insieme i 150 anni di vita. Assistiamo oggi ad un rinnovato amore dei cittadini verso il proprio Paese, verso la nostra patria. Le sempre più presenti espressioni politiche che ne mettono in evidenza i caratteri regionali e territoriali non fanno altro che esaltarne le diversità nell'unità, le ricchezze nazionali e nello stesso tempo le necessità locali. La nostra è sempre stata una terra di grandi talenti, dove sono nati ed hanno operato geni che hanno fatto la storia dell'umanità. Dobbiamo dunque rafforzare nel mondo l'immagine di un'Italia che produce, che crea, che esporta, che è orgogliosa della propria storia e delle proprie tradizioni e che, davanti alle difficoltà, sa reagire con determinazione. Lo dimostrano le decine di migliaia di imprenditori che, nonostante le oggettive difficoltà della congiuntura internazionale, riescono a tenere testa alla sfida globale. Dobbiamo difendere senza tentennamenti le nostre radici cristiane, la nostra identità che tanto ha contribuito alla nascita dell'Occidente e della nostra civiltà. Dimenticare le proprie radici significa perdere l'anima, non ritrovare più se stessi, non trovare più le ragioni forti dell'appartenenza che ci permettono di accogliere e dialogare con gli altri senza cedimenti e senza ipocrisie. L'Occidente, l'Europa e l'Italia o ritornano alle proprie radici o sono destinati ad un irreversibile tramonto. Siamo chiamati dunque a tenere alto il nome ed il prestigio dell'Italia, sia nel contesto dell'Europa unita, di cui siamo stati fin dall'inizio fondatori, sia nel contesto internazionale, attraverso il saldo rapporto atlantico ed il ruolo geopolitico nella grande area del Mediterraneo. Il nostro Paese deve ribadire sempre di più al mondo il suo ruolo di portatore di pace e di democrazia. Sulla concreta solidarietà democratica ai Paesi in difficoltà l'Italia sta offrendo un contributo di altissimo valore. Ha il merito, che nasce da un dovere umanitario, delle missioni di pace che sotto l'egida dell'ONU contribuiscono all'impianto di servizi umanitari e spesso all'avviamento di nuove democrazie. Seguiamo con ammirazione e partecipazione l'operato dei nostri uomini impegnati in questi rischiosi territori e a loro va la nostra sincera gratitudine. Il nostro pensiero gratissimo e commosso va anche a coloro che hanno sacrificato la vita per l'umanità in nome dell'Italia e dei suoi valori: ai ragazzi di Nasiriya e agli altri che, come loro, hanno scritto il loro nome nel Pantheon degli eroi della pace.

ricordo, quello di questi uomini caduti per la pace, che rimane indissolubilmente congiunto ad un altro: al ricordo della compostezza con cui i loro cari hanno vissuto la loro tragedia familiare. È stata una vera, indimenticabile lezione per tutti. Voglio rivolgere un pensiero a quegli eroi civili della lotta alla mafia che, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, hanno donato la loro intelligenza e la loro

troppi caduti tra magistrati, uomini delle forze dell'ordine, giornalisti, imprenditori ai quali ci inchiniamo, riconoscenti e debitori. Di grande consolazione e certo non di rassegnazione appare a tutti l'evidente spinta che li ha mossi a difendere i nostri valori più importanti, quella cioè di preservare dalla violenza e dalla oppressione criminale il nostro futuro, il futuro dei nostri figli. È proprio a loro, ai giovani, a quelli cui siamo chiamati a consegnare un'Italia più florida e più sana che voglio dedicare il mio pensiero conclusivo. Ai giovani chiediamo di guardare alla politica e alla forza delle istituzioni, perché alle loro istanze, che sappiamo essere prioritariamente la casa, il lavoro e la cultura, risponderemo con l'impegno e l'ausilio necessario di tutte le forze politiche. La nostra saggezza - se c'è - vale come testimonianza e patrimonio per la loro audacia, il loro entusiasmo e la loro fiducia. Siamo chiamati a sostenerli nel percorso che li porta a diventare adulti e a svolgere i ruoli che oggi noi svolgiamo. Soltanto se avremo le carte in regola, se avremo fatto quanto dovuto e quanto necessario, potremo guardarli negli occhi e vedere rispecchiato il nostro Paese, la nostra Italia. Viva il Senato, viva l'Italia!

Prego gli onorevoli colleghi di voler prestare attenzione alle seguenti comunicazioni. Ricordo che, a norma dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento, entro le ore 13 di venerdì 2 maggio, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, i Gruppi parlamentari sono convocati per lunedì 5 maggio alle ore 18, per procedere, ove non lo avessero fatto in precedenza, alla propria costituzione.

per l'elezione dei quattro Vice Presidenti, dei tre senatori Questori e degli otto senatori Segretari». La seduta è tolta *(ore